un uomo, un atleta italiano, un ragazzo del Sud nato in Puglia nella mia città, Barletta, e conosciuto in tutto il mondo per le sue straordinarie imprese sportive. Sto parlando del compianto Pietro Mennea, scomparso prematuramente a soli sessant'anni proprio il 21 marzo di sei anni fa, nel 2013. Pietro Mennea è una leggenda dello sport mondiale, un uomo prima che un atleta per tutti simbolo di forza di volontà e tenacia oltre ogni limite, oltre la fatica, oltre i limiti fisici, oltre la sofferenza. Non a caso amava ripetere sempre le parole: «soffri ma sogni» per esprimere la dimensione totalizzante del suo impegno, della sua determinazione a inseguire un obiettivo che per tutti poteva sembrare solo un sogno, ma che lui ha saputo tramutare in straordinaria realtà di vita. Pietro Mennea negli anni Settanta e Ottanta è stato il simbolo dell'Italia e soprattutto di quel Sud che cerca di trovare riscatto attraverso l'impegno e la volontà di affermarsi con le proprie forze; un ragazzo non particolarmente dotato fisicamente che sfida i muscoli delle potenze mondiali, come Unione Sovietica e Stati Uniti, e vince sospinto dal vento del suo inarrestabile sogno. A soli vent'anni nel 1972 partecipa già alle prime Olimpiadi e si classifica terzo nei 200 metri, dopo Borzov e Larry Black, che erano dei giganti in quel momento. Il 1979 (e quest'anno ricorrono anche i quarant'anni del *record* del mondo) è l'anno d'oro di Pietro Mennea, che da studente universitario partecipa

e 72), che sono una pietra miliare dello sport italiano. Mennea confermerà poi la sua supremazia anche a Barletta con un tempo di 19 secondi e 96 centesimi; nel 1980 raggiunge anche l'apice perché vince la medaglia d'oro a Mosca e tutti nella nostra memoria ricordiamo quella gara, anche quella storica ed epica. Oramai Mennea viene conosciuto in tutto il mondo come la "freccia del Sud", ma proprio all'apice del suo trionfo decide di smettere, di dedicarsi alla sua vita,

Vorremmo che fosse ricordato dalle nuove generazioni che non hanno avuto come noi la fortuna di seguire in diretta le sue imprese di quegli anni. Non importa quali siano le condizioni di partenza, ciò che conta è la grinta che si è capaci di tirare fuori nel percorso, che sia una pista d'atletica o la vita quotidiana.

*(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi onora in questa giornata e in questo luogo ricordare la memoria del grande atleta Pietro Mennea, campione e cittadino della città di Barletta. Mi piace ricordarlo, perché i valori dello sport sono comunque valori esistenziali che devono continuare a mantenere saldi i valori umani. È importante ricordarlo in questo giorno per l'impegno, anche politico, esercitato da grande campione. Pietro Mennea continua ad essere un baluardo e soprattutto un paradigma di comportamento per le giovani generazioni e per tutti noi che ancora guardiamo con attenzione ai valori etici e morali della nostra pratica politica. Ringrazio tutti i colleghi che in questo momento si sono senz'altro uniti a me in questo ricordo, perché esso possa essere comunque un elemento di prospettiva e, soprattutto, possa indicare una strada netta, tersa e compiuta di responsabilità in qualsiasi ambito e in qualsiasi luogo. Vi ringrazio per l'attenzione nel ricordo di Pietro Mennea, campione e cittadino della città di Barletta. Grazie!

sabato scorso a Roma c'è stata una grande manifestazione del settore dell'edilizia. Imprese, sindacati, operai, lavoratori del settore, professionisti: 15.000 persone in piazza per manifestare la difficoltà economica di un settore importante per l'economia italiana. Un settore che negli ultimi anni, dall'inizio della crisi, ha visto perdersi 600.000 posti di lavoro, 120.000 imprese chiudere e due delle tre principali imprese italiane per fatturato, importantissimi gruppi che hanno tenuto alto il nome dell'ingegneria italiana nel mondo, in gravissima crisi, a un passo dalla chiusura. I dati dell'economia sono noti a tutti. È stata fatta una legge di bilancio bluffando sui numeri, non solo solo sopravvalutando il segno "più", ma negando che rischiamo di avere segni "meno" quanto a prodotto interno lordo. In questo quadro, un Governo serio, che sia sul pezzo, che voglia guardare allo sviluppo del Paese, investe nel settore delle costruzioni. Qualsiasi economista sa che è il settore che dà in più breve tempo la risposta più veloce: si dice, tipicamente, anticiclica. Leggiamo sul giornale di oggi e nei giorni scorsi dello sblocca cantieri; lo leggeremo. Per ora vediamo soltanto una polemica, l'ennesima, tra due forze politiche che, fino alle elezioni europee di maggio, probabilmente non riusciranno a a varare nessuna misura e troveranno gli accordi soltanto su vicende che poco hanno a che fare con la politica, come quella a cui abbiamo assistito ieri in Parlamento: un accordo netto tra MoVimento e Lega, che probabilmente sarà ripetuto stamattina, e non vogliamo pensare che la quasi coincidenza di date abbia una motivazione maliziosa. Lo sblocca cantieri che cosa sarà? Vedremo. Adesso sembra che ci sia un braccio di ferro per capire se si possa o no infilare l'ennesimo condono più o meno mascherato. Qualcuno pensa che le opere pubbliche riprendano perché cambiano le leggi, perché si fa diminuire la soglia di trasparenza, perché si rende più facile la corruzione velocizzando l'*iter* delle procedure? Non è così. Nell'ultima audizione che abbiamo avuto in Commissione, l'audizione di Invitalia (la più grande centrale di committenza), ci è stato detto che, a codice degli appalti vigente, quella centrale di committenza ha appaltato 272 opere con il contenzioso, e soltanto nel 7 opere sono partite. Il problema, quindi, non è il codice, ma avere pubbliche amministrazioni e stazioni appaltanti che sappiano fare il proprio lavoro e - ancora di più - soldi più - soldi da investire. Tuttavia, se nella legge di bilancio i soldi vengono destinati non allo sviluppo, all'impresa e all'economia, ma ad altre misure come il reddito di cittadinanza e quota 100, si fa una scelta politica chiara e rispettabile, secondo me completamente contraria alle

La mozione è sostanzialmente incentrata, ancora una volta, su un balletto - questa volta ancora più indecoroso - relativo alla TAV. Potrei svolgere sull'argomento tantissime considerazioni, perché l'intera procedura seguita fa acqua da tutte le parti. Seguiamo un ordine cronologico inverso.

Si inventa una strana procedura, o - meglio - una procedura ordinaria la si fa diventare straordinaria. Mi riferisco alla clausola di dissolvenza inserita nel bando, che poi, usando la terminologia francese, si chiama avviso preliminare.

l'ultima clamorosa figuraccia che abbiamo fatto come Paese, perché poi le cose ce le diciamo qui, ma credo che di noi ridano un po' dappertutto nell'Unione europea per la soluzione individuata. Se andiamo *ab origine*, la serie di perle inanellate nella costruzione di questa procedura da parte del ministro Toninelli è infinita. Si parla dell'analisi costi-benefici come se fosse un'invenzione e diventa un mantra. Tutti - o almeno gli operatori del settore - sanno che l'analisi costi-benefici è un'altra cosa ordinaria da almeno vent'anni, peraltro resa obbligatoria dalla tanto vituperata - magari erroneamente - legge obiettivo. Su quest'opera l'analisi costi-benefici è stata ripetuta più volte in maniera molto rigorosa. Sembra che questo Governo abbia scoperto l'analisi costi-benefici. Poi scopriamo - ma lo avevamo detto un anno fa - che non è altro che un espediente per prendere tempo e se avessero potuto prenderne altro due settimane fa, lo avrebbero fatto. ripeto, le perle inanellate sono tantissime. Anche in questo caso, partiamo dall'ultima. Sembra una barzelletta, ma - purtroppo - non lo è. Anche questa non ci fa fare bella figura nel Paese. Il Presidente della commissione che ha redatto l'analisi costi-benefici, professor Ponti (in questo caso non *nomen omen*),

europea un documento in cui si dice che l'opera va bene. Quindi, con una mano in Italia dice che l'opera «non s'ha da fare» e con l'altra, invece, la propria società viene pagata in maniera sufficientemente vantaggiosa per dire che l'opera va bene.

Si prendono "x-1" commissari, che già avevano scritto in tutto il mondo documenti contro la TAV, più un commissario che, invece, era neutrale all'inizio del lavoro e si costituisce una commissione di fare l'analisi costi-benefici. Insomma, come ho detto in un'altra circostanza, Totò direbbe che si è data la traccia: cari, prendete molto tempo, scrivete alla fine che l'analisi costi-benefici non funziona perché noi quest'opera la dobbiamo bloccare per prendere un po' di applausi da parte dei No TAV. L'inganno è venuto immediatamente fuori: l'ingegner Coppola non ha firmato l'analisi costi-benefici; dopo la consegna, lo stesso presidente del Consiglio Conte ha chiesto di rivederla perché c'era un errore marchiano. Ha detto che si trattava di un errore grossolano da correggere: "ballavano" un paio di miliardi di euro. Questa analisi costi-benefici non sta in piedi; considera un beneficio ambientale come un costo: costruire la TAV significa far camminare meno macchine e tir lungo la strada quindi, consumare meno benzina - cosa che dovrebbe essere una scelta politica di ogni Governo, come lo è stata per il Partito Democratico, che sulla cura del ferro ha investito *(Applausi dal Gruppo PD)* - e, invece, diventa un maleficio perché diminuiscono le accise della benzina.

giusto che il Senato votasse la sfiducia al ministro Toninelli per molta incompetenza, per grande incoerenza e per il fatto di danneggiare gravemente l'economia del nostro Paese. Grazie!

una mozione di sfiducia individuale. Vorrei spiegarvi perché Forza Italia nella sua venticinquennale storia parlamentare ha deciso di prendere una posizione così distante dal suo naturale sentire politico. sentire politico. Ministro Toninelli, il suo caso è un *unicum*. Ministro Toninelli, noi non ce l'abbiamo con lei. Ministro Toninelli, non è colpa sua. Noi comprendiamo bene che essere Toninelli oggi è una condizione pesante Noi siamo assolutamente solidali con lei da questo punto di vista perché lei non ha bisogno di nemici o di detrattori perché lei è il miglior detrattore di se stesso ed è bravissimo a fare tutto da solo. Ogni giorno un italiano si sveglia e sa che prima di sera arriverà una *gaffe* del ministro Toninelli. Ci sarebbe da sorridere se le sue fossero le battute comiche da cui è partito il MoVimento 5 Stelle e, invece, non sono battute e, quindi, non c'è proprio niente da ridere. Non si può scherzare sulla pelle degli italiani e dell'Italia sulla perdita di migliaia di posti di lavoro. Non si può scherzare sulla reputazione di un Paese intero. Non si può scherzare sulla credibilità del nostro Governo all'estero e in Europa. Non si può scherzare sui soldi dei contribuenti; non si può scherzare sul futuro dei nostri figli. C'è da stare seri più che mai perché il problema è serio. Il problema forse è anche la leggerezza con cui lei ha accettato di ricoprire un ruolo così impegnativo e strategico per la vita di una Nazione come l'Italia senza forse comprenderne appieno le implicazioni e l'incredibile responsabilità. Questo la dice lunga sulla sua capacità di consapevolezza. Partecipare al Governo di un Paese non è come partecipare al programma "la Corrida" di Corrado. Sarebbe come se a me, se a me, dilettante assoluta del tennis, mettessero la racchetta in mano per sfidare Federer in Coppa Davis per rappresentare l'Italia. *(Applausi oltre la follia, come scrive lei in uno dei suoi ultimi *post* su Facebook - perché si parla attraverso i *post* di Facebook - con riferimento al fatto che dei matti la criticano perché promuove le auto elettriche e compra l'auto *diesel*. Ora, il problema, ministro Toninelli, è dove ha intenzione di portare l'Italia e gli italiani con le sue non scelte dissennate, dove lei ha intenzione di portare l'Italia con il suo atteggiamento superficiale, con le sue esternazioni agghiaccianti e i comportamenti irrispettosi. Come quella volta quando il collega Biasotti, rievocando la tragedia del ponte Morandi di Genova con le lacrime agli occhi, si rivolgeva a lei, Ministro, che rimase per tutto il tempo con la testa bassa e gli occhi fissi sul cellulare e ai richiami dell'Assemblea rispondeva si ascolta con le orecchie mentre una classe di studenti assisteva. Noi lo sappiamo dove lei, ministro Toninelli, ha intenzione di portare l'Italia: lei ha intenzione di portare l'Italia dentro un *tunnel* in fondo al quale, però, è in arrivo un treno ad alta velocità e il Paese tutto ci va a sbattere. Il problema, quindi, è serio, molto serio, e noi, contro ogni inclinazione che ci è naturale come forza politica liberale e garantista, come forza politica che fa del sì il suo *slogan* ricorrente, oggi le diciamo un grande, secco, sonoro, fortissimo no! No, perché il nostro dovere è prima di tutto quello di salvaguardare la nostra Nazione, di provare con tutte le nostre forze a reinnestare la marcia per farlo ripartire, per tirarlo fuori dalla palude finché ancora il naso è fuori e riesce a respirare, fuori dalla stagnazione prima che si trasformi in recessione irreversibile. La decrescita felice non è la condizione naturale per l'Italia e per il suo popolo, per un Paese che ha una posizione strategica all'interno del Mediterraneo. Quello che ci atterrisce è la totale mancanza di visione strategica, di cosa vuol fare da grande questa Nazione. Quello che ci atterrisce è l'improvvisazione che, seguendo la sua vocazione naturale, Ministro, quella che dovrebbe seguire,

è che non è che scegliendo di non completare la TAV, per citare il caso più eclatante, il resto dell'Europa si ferma. La TAV non è solo il pezzettino che passa per l'Italia,

risultato è che diventeremo una boa. Avete presente una boa? Provate a immaginare l'Italia come la boa delle regate, ferma in mezzo al mare, galleggiante, paciosa, con tutte le barche che sfrecciano velocissime intorno a lei, in competizione per la vittoria, stando bene attenti a non toccarla, la boa, pena la squalifica. No, ministro Toninelli, non è questo che il nostro Paese si merita: il Paese che con tre caravelle è andato a scoprire l'America, ora rischia di diventare una boa in mezzo al mar Mediterraneo. No! *(Applausi dal Gruppo La beffa della TAV è che comunque la quota di fondi spettante all'Italia la dovremo pagare lo stesso. E quindi cosa dovremmo dirle, ministro Toninelli, per questo regalino GALLONE *(FI-BP)*. Cosa le dovremmo dire per questo regalino che vorrebbe fare ad un Paese che ha già un debito pubblico esorbitante? Dovremmo dirle: «Grazie per volerci impoverire ancora di più»? Dovremmo dirle: «Grazie per le scelte che vorrebbe compiere nonostante noi e con i soldi degli italiani?». No, le diciamo «no, grazie», perché non vogliamo passare dal decreto sblocca cantieri, che è solo un titolo ad effetto, al blocco al blocco dell'Italia, come anche gli alleati della Lega temono. Oggi è scritto a chiare lettere sui giornali; il *premier* Conte nel corso del suo intervento sulla cosiddetta Via Via della Seta (altro nome evocativo e affascinante, che nasconde pericoli se non declinato e attuato con attenzione e competenza estrema se non vogliamo che accada quanto accaduto agli Stati Uniti) agli Stati Uniti) ha parlato di diversi corridoi strategici. Invece noi rischieremo anche di vederci passare i *container* che duplicheranno, dopo il raddoppio del Canale di Suez, sopra la testa, verso Rotterdam, verso l'Olanda. Visualizziamo sempre la boa.

Noi oggi con la mozione di sfiducia nei suoi confronti dimostriamo di esserle amici, di volerle dare un *assist* importante. Tiri lei il calcio della vittoria; visualizzi la porta, si dimetta e faccia vincere il Paese. Ministro Toninelli, lo facciamo per lei.

anche se l'esito mi sembra del tutto scontato. Vorrei dire peraltro che sulla delegittimazione del Ministro si sono lette tante cose in queste ore e nelle settimane scorse. Non so e non sappiamo come sarà il decreto

sul clima che le propongono le opposizioni, ma su quello che trova dentro la stessa maggioranza.

Il problema di come il Governo - e lei, oggettivamente, in quanto responsabile del Dicastero - sta gestendo questa vicenda è, per alcuni aspetti, veramente incredibile. onde evitare di assumere una decisione si usano gli espedienti che, agli occhi di tutta l'Europa, risultano e risulteranno sempre più ridicoli.

Su questo dovreste avere il coraggio di decidere; non ce l'avete, aspettate il 26 maggio, ci sono le elezioni, ciascuno deve dire che ha vinto, che va avanti la propria tesi. È davvero una presa in giro per gli italiani. Il problema è che a pagarne il conto è l'Italia, un Paese in recessione, un Paese in grave difficoltà economica che, oggettivamente, vede la fine del 2019 e l'elaborazione della legge di bilancio per il 2020 come un ostacolo veramente altissimo. Dunque, il livello di

Aggiungo un'ultima questione, Ministro. Ciò che più mi colpisce, oltre alla vicenda della linea TAV, è che è passato ormai un anno: non si comprende qual è la strategia, qual è la programmazione, che cosa si intenda fare. Non si capisce dove il Governo intenda agire - realmente, non con le dichiarazioni e la propaganda - per portare questo Paese ad un salto indispensabile dal punto di vista infrastrutturale. Tutte le volte che si discute di un'opera, alla fine troviamo, nel territorio prima, e nel dibattito in seno al Governo poi, una dialettica che tiene bloccato tutto. Questo è un grandissimo problema. Ministro, lei dovrebbe assumersi la responsabilità, a partire da questo dibattito, di dire

Signor Presidente, dopo aver ascoltato l'illustrazione del documento che il mio Gruppo pone oggi all'attenzione dell'Assemblea, emerge, con amara nitidezza, una considerazione che scavalca ogni discussione di merito e di cui anche i proponenti - dire compreso il sottoscritto - devono prendere coscienza. Dobbiamo prendere coscienza che il ministro Toninelli è già sfiduciato nei fatti, e un voto contrario alla mozione del Partito Democratico nient'altro sarebbe che negare la verità storica di una parabola discendente che ha condotto il responsabile delle infrastrutture e dei trasporti a perdere qualsivoglia credibilità di fronte ai nostri concittadini, al tessuto produttivo e alla comunità internazionale rappresentata dalle istituzioni europee. Lo abbiamo sentito oggi nella disamina del collega Margiotta; lo abbiamo letto per mesi sui giornali e sul *web*; lo abbiamo ascoltato nelle parole di esperti, centri di ricerca e organismi imparziali. Le vicende che hanno interessato la gestione del progetto Alta Velocità Torino-Lione dall'inizio della legislatura costituiscono, di per sé stesse, una sentenza di condanna dell'operato del ministro Toninelli e sono la rappresentazione plastica di come il Ministro stia affrontando tutto il tema delle infrastrutture del nostro Paese. Per quanto riguarda la strategica infrastruttura Torino-Lione, eravamo partiti dalla nuova analisi del rapporto tra costi e benefici, una chimera cui nemmeno il Ministro ha mai creduto davvero e che, alla fine, si è rivelata un *boomerang* anche per chi nell'Esecutivo se ne è servito con l'intenzione di prendere tempo. Si andava cercando una pezza d'appoggio per giustificare un altrimenti scomodo disimpegno dell'Italia nella realizzazione dell'opera. Ma nemmeno i plurimi tentativi di manipolazione dei dati e di mistificazione della lettura hanno sortito l'effetto sperato dal Ministro, tanto che persino il *premier* Conte ha tentato di mettere in atto dei disperati aggiustamenti. Così è cominciata la strategia suicida che ci ha condotto fin sulla soglia dell'ipotesi di un mini TAV, che per il Nord Ovest e per il Piemonte significherebbe esattamente essere tagliati fuori dalla tratta ferroviaria e dalle sue positive ricadute in termini di sviluppo economico. Nel mentre, si è affacciato il rischio di dover rinunciare ai finanziamenti europei e, in assenza di certezze, politiche soprattutto, e di una guida salda, ha prevalso, di nuovo, la logica del temporeggiatore. Ma con la clausola di dissolvenza a pagare l'incertezza saranno, innanzitutto, le imprese. La narrazione sulla clausola di dissolvenza, cioè questo straordinario espediente giuridico previsto dall'ordinamento francese, è servito a rassicurare solo gli elettori del MoVimento 5 Stelle. Caro Ministro, lei ha il dovere di spiegare agli italiani che anche nel nostro ordinamento è prevista la facoltà per le stazioni appaltanti di interrompere la procedura di gara in presenza di nuovi elementi ostativi. Con questa verità, però, non avrebbe potuto rassicurare

La sentenza di condanna dell'operato ministeriale, colleghe e colleghi, allora è già scritta e questa Assemblea ha il dovere di ratificarla, se non vuol fare la fine dell'ultimo giapponese. Certifichiamo il fallimento, che è già sotto gli occhi di tutti, e poniamo termine alla guerra delle contraddizioni e delle mistificazioni della realtà addomesticata, per poter almeno sperare ancora in un cambio di passo e per ridare al Paese la reputazione necessaria a trattare con gli interlocutori del progetto, pubblico e privato.

che, nell'incertezza, si è reso strategicamente complice. Il destino è dell'Italia, della sua economia nazionale e internazionale. L'unico destino di cui dovrebbe importarci.

esclusivamente sulla vicenda TAV, che non si dovrebbero preoccupare. Non so perché vi state così preoccupando, perché ho l'impressione che, con tutta la sceneggiata che è stata messa in atto sulla vicenda dei bandi che partono e non partono e la clausola di dissolvenza, come tutti sappiamo, si cerca solo di prendere tempo.

io sono stata prima firmataria di un ordine del giorno che le chiedeva di assumere una decisione chiara,

alla vicenda della linea TAV, perché la consideriamo un'opera assolutamente inutile e dannosa. D'altronde, se per vent'anni non s'è fatta, qualcuno mi dovrà dare una spiegazione. Per quanto mi riguarda,

Evidentemente il contratto di Governo è solo e costantemente declinato sugli assi e i voleri della Lega stessa. Confermo il fatto che

Va detto in questo caso che certamente il ministro Toninelli è passato agli onori della cronaca più che per le azioni positive o anche negative del suo Dicastero,

con altro nome, magari più fantasioso, la "delega del futuro": le infrastrutture di una Nazione attengono strettamente alla sua capacità di stare dentro il futuro e intercettare il progresso.

si insediò, aveva sul tavolo lavori per circa 23 miliardi di euro, che cerco brevemente di riepilogare: il Terzo valico dei Giovi lungo l'asse Genova-Milano, per un valore globale di 6,2 miliardi, bloccati dall'analisi costi-benefici della famosa commissione del professor Ponti; l'asse Brescia-Verona, approvata dal CIPE, per 2 miliardi di euro, con atto integrativo firmato da Rete ferroviaria italiana con il g*eneral contractor*, bloccata anche questa dalla famosa commissione del professor Ponti; l'asse Verona-Bivio Vicenza, opera approvata dal CIPE per un importo di 2,7 di 2,7 miliardi, per cui è in corso la sottoscrizione dell'atto integrativo di Rete ferroviaria italiana e del *general contractor*, ma anche in questo caso l'opera è bloccata dalla commissione del professor Ponti. la Vicenza-Padova, progetto definitivo disponibile, compreso il nodo di Vicenza: non c'è bisogno di fare la gara, esiste apposita concessione al *general contractor*, ma anche in questo caso l'opera è bloccata dal mitico professor

attualmente sono stati affidati due lotti per un importo globale di circa 700 milioni euro, la parte restante è di 3,4 miliardi di euro e il commissario, attualmente amministratore delegato di Rete ferroviaria italiana, potrebbe affidare i vari lotti utilizzando modalità che trasferiscono ai vincitori delle gare anche la redazione dei progetti. Per l'asse Palermo-Catania l'importo dell'opera si attesta su un valore pari a 5 miliardi di euro per la realizzazione degli interventi è previsto apposito commissario straordinario con pieni poteri; attualmente è escluso il primo lotto nella zona di Himera e non è stato affidato nulla. Anche in quest'ultimo caso il commissario è l'attuale amministratore di Rete ferroviaria italiana: potrebbe affidare i lotti utilizzando le modalità che trasferiscono, di cui sopra. Da questo elenco,

quanto avete fatto con l'ultima finanziaria, e cioè il taglio a Rete ferroviaria italiana di 2,6 miliardi di euro che blocca praticamente ogni attività per tutto il 2019, analogamente l'avete fatto per tutte le opere che ho appena

che cosa avete fatto di quelle risorse? Ce lo dice, Ministro? Vede, rispetto alle parole per le quali lei è passato alla storia, noi registriamo anche la vicenda dello smontaggio della fusione tra Anas e Ferrovie

davanti alle parole dello Stato, la gente si fida, tende ancora a fidarsi, nonostante tutto; le aziende fanno i loro progetti e le amministrazioni locali decidono il loro piano di investimenti.

i decisori, i gestori e i consigli di amministrazione aspettano di capire che cosa succede. Dobbiamo rismontare questa fusione? Ce lo dica, Ministro, perché non basta declamare,

della Astaldi e quanto sta accadendo con un numero enorme di imprese che stanno saltando come le castagne sul fuoco. Quelle imprese hanno lavorato, signor

- non siamo affascinati più di tanto dalle mozioni di sfiducia individuale, anche perché credo che i numeri dell'Assemblea

Che cosa sta succedendo all'interno dell'importantissima delega delle infrastrutture? L'infrastrutturazione dell'Italia sconta un *gap* drammatico che deve rapidamente essere colmato. Fate quello che volete, ma fate

per giustificare la sfiducia nei confronti del ministro Toninelli basterebbe solo ricordare che è l'unico Ministro delle che, nell'anno in cui è stato in carica, più o meno, non solo non ha avviato alcuna opera fondamentale per il nostro Paese, ma addirittura sta facendo di tutto per bloccare tutte quelle che erano state previste nel passato. *(Applausi dal Gruppo PD)*. In altre Nazioni credo che lo avrebbero già cacciato via. In ogni caso ci sono almeno sei buone ragioni per la sfiducia al Ministro. La prima è che in tutti i Paesi, come anche in Italia, la velocità della ripresa economica e la competitività e la competitività dipendono in buona parte dagli investimenti, dalle grandi opere infrastrutturali, cioè dalla capacità di guardare al futuro e dotare il Paese di infrastrutture per cogliere Al contrario, invece, in Italia la decisione che il Ministro ha assunto è bloccare quasi tutte le opere, addirittura quelle in corso di realizzazione, alcune delle quali già in parte finanziate. È un qualcosa di clamoroso che mette in difficoltà le imprese, i lavoratori, lo sviluppo del Paese e compromette gli accordi che l'Italia ha stipulato in sede europea. Lei è responsabile, signor Ministro, della paralisi infrastrutturale che deriva dalla sua scelta infelice di nominare un gruppo di contrari a tutto un incarico che ha a che vedere con lo sviluppo dell'Italia. Lei ha operato scientemente per impedirlo, addirittura intervenendo più volte per orientare in senso negativo le conclusioni di quel gruppo. Inoltre, ha dimostrato palese inadeguatezza: i suoi annunci sui tempi delle conclusioni delle analisi costi-benefici sono sempre stati fasulli. Lei ha giocato sulla pelle dell'Italia; ha portato avanti la sua visione negativa dello sviluppo; è arrivato al punto di consentire l'inserimento tutto in quell'analisi: per capirci, mancava solo il costo dei rifiuti che i lavoratori produrranno durante la realizzazione delle opere per completare le assurdità contenute in quell'analisi. Lei ha sottratto ogni informazione al Parlamento: i dati li abbiamo conosciuti dalla stampa, mai dal suo Ministero e, peraltro, sono membro della Commissione competente. Abbiamo letto quei dati dalla stampa. Se non ricordo male, lei professava trasparenza in occasione dell'esame delle mozioni alla Camera, ma si è qualificato con un comportamento omertoso, che ha a che vedere con una visione proprietaria del bene pubblico. Lei ha esposto il Paese a contraddizioni e contrasti con altri Paesi europei. Su molti degli accordi lei ha isolato l'Italia. Siamo isolati; la collega prima intervenuta parlava di boa e immagino

Caro Ministro della decrescita felice *(Applausi dal Gruppo PD)*, noi non vogliamo un Paese che torni al Medioevo; anzi, le abbiamo lasciato un'eredità importante, miliardi di euro e progetti (connettere l'Italia, la cura del ferro), ma lei sta facendo di tutto per destrutturare Noi siamo convinti che la prospettiva dell'Italia sia nella crescita e nello sviluppo e che per perseguirla, e quindi per il bene dell'Italia, sia più che opportuno che lei lasci l'incarico, perché sta smantellando tutto. Io penso che nessun italiano si lamenterà della sua assenza se lei non è al

la sfiducia al ministro Toninelli. Il richiamo esclusivo al motivo TAV è oltremodo limitante e divisivo. In effetti, il ministro Toninelli ha ben altri motivi per dimettersi, molto più gravi. Il ministro Toninelli si dovrebbe dimettere - secondo me - perché è stato sostanzialmente assente dai suoi specifici compiti e ha lasciato la gestione della portualità e delle vicende connesse con i naufragi alla incompetenza del ministro Salvini.

si è potuta creare per la totale assenza di intervento del soggetto posto a capo dell'Amministrazione responsabile anche dello sbarco. Ieri ne abbiamo parlato: anche dello sbarco in porto è responsabile l'Amministrazione marittima. anche dello sbarco in porto è responsabile l'Amministrazione marittima. Viceversa, dell'immigrazione è responsabile l'altro Ministro; ma lo sbarco in porto, l'approdo di naufraghi è responsabilità dell'Amministrazione marittima, e il Ministro ha latitato. Sì, c'è una paralisi infrastrutturale, c'è una latitanza. Ecco il motivo per il quale io voterò comunque la sfiducia, nonostante le vostre proposte limitate e divisive.

abbiamo esitato un po' quando abbiamo pensato di presentare la mozione di sfiducia, ma non per i termini che ricordava il collega De Falco. Francamente, sul piano politico, più lei rimane a fare il Ministro e più *chance* abbiamo noi di vincere le prossime elezioni europee. È evidente che l'interesse dei cittadini ha prevalso su questo interesse politico e, quindi, abbiamo pensato, avendo elementi più che sufficienti, di presentarla ugualmente. Qualche cosa l'avevamo capita già dal suo insediamento. Io sono membro della Commissione trasporti, lavori pubblici e comunicazione del Senato

quando tutti i Ministri del vostro Governo si sono recati alle Commissioni parlamentari per l'indirizzo di mandato dopo pochi giorni dall'insediamento del Governo, lei se ne è ben guardato ed è arrivato non prima del 31 luglio, con due mesi di ritardo, tenendo di fatto in ostaggio la Commissione che non sapeva tecnicamente quello che lei aveva in mente di fare.

quando poi si è presentato, il 31 luglio dello scorso anno (quindi con due mesi di ritardo), abbiamo scoperto - lo dico ai rappresentanti della maggioranza - quello che lei aveva in mente che le opere pubbliche in generale fossero un problema per lei, che rappresenta appieno il MoVimento 5 Stelle. Io dico tante volte che il MoVimento 5 Stelle è coerente da questo punto di vista,

Non so se ricorda la battuta che feci al presidente Schifani, che sedeva affianco a me in Commissione in quella occasione. Dissi che il problema è particolare per il presidente Schifani perché, venendo da Palermo, in bicicletta arriva al massimo a Messina e non riuscirà neanche a passare

rilevato che le opere bloccate sono più di 28 e riguardano tutte le Regioni. Io vivo in Toscana e le ricordo la terza corsia tra Firenze e Pistoia, l'autostrada tirrenica e il sistema della tangenziale lucchese. Peraltro, sulla questione degli assi viari ancora non ci è dato sapere quello che lei ha nella testa

detto che il suo è il «Ministero del viaggio» e che «nulla più del viaggio può far crescere, progredire, migliorare e, in definitiva, può far sognare tante persone».

su cui spenderei un minuto. Lei, Ministro, ha bloccato addirittura il piano industriale approvato nel 2018, altrimenti i controllori di volo avrebbero scioperato. Ma le ricordo che il 57 per cento della proprietà dell'ENAV è dello Stato e lei lo deve gestire, Ministro. Si faccia un appuntino: scriva ENAV da una parte. E meno male che vi hanno fermato su Fincantieri e affini, ma perché sono intervenuti i mercati internazionali, altrimenti nessuno

ha investito settimane e ancora stiamo facendo audizioni sulla questione del codice degli appalti. A un certo punto, una mattina - ho posto la questione ufficialmente in Commissione - scopriamo, tramite il nostro Ufficio studi, di aver ricevuto una velina della legge delega sul codice degli appalti con una definizione di dettaglio di quello che sarebbe stato il futuro della legge sul codice degli appalti. Il Parlamento sapete dove è? Il Parlamento avrà il diritto di decidere qualcosa sulla questione del codice degli appalti, oppure facciamo l'errore della precedente legislatura quando abbiamo delegato un magistrato e l'ANAC a fare un codice degli appalti che ha messo in ginocchio il nostro Paese? Mi sta lampeggiando il microfono e ciò significa che siamo arrivati alla fine dell'intervento. Ministro, voglio dirle

espressi contro la mozione di sfiducia, visto che ieri la maggioranza ne ha espressi soltanto 153 per salvare il signor ministro dell'interno, senatore Salvini, e sono stati necessari i nostri voti per evitare che il ministro Salvini andasse sotto processo. Oggi voglio vedere se saranno più di 153 i voti che salveranno lei, perché il suo Gruppo ha fatto mancare l'appoggio a quella maggioranza che avrebbe mandato sotto processo un uomo che ha difeso l'interesse dello Stato. Dichiaro chiusa la discussione. Ha chiesto di intervenire il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, senatore Toninelli. trasporti*. Presidente, colleghi, voglio ringraziare coloro i quali con le mozioni in esame mi danno la possibilità di raccontare il lavoro fatto nei nove mesi di Governo. La prima importante questione che ci siamo trovati ad affrontare in estate è stata l'ondata migratoria nel Mediterraneo. Lo abbiamo fatto nel rispetto dei diritti umani, ma finalmente anche applicando la fermezza necessaria per il ripristino della legalità e delle convenzioni internazionali. Grazie al lavoro del Governo il numero dei barconi della morte salpati dalla Libia è diminuito drasticamente nell'ultimo anno. Cito solo il dato significativo del primo scorcio del 2019: dal 1° gennaio al 20 marzo sono stati soccorsi 398 migranti contro i 6.161 dello stesso periodo del 2018, un calo del 94 per cento, con una Guardia costiera

una buona notizia che non basta, ovviamente, perché vogliamo azzerare del tutto questi numeri, ma i primi mesi di azione di questo Governo sono più che incoraggianti. Per la prima volta, grazie al nostro operato, sono state realmente poste al centro del dibattito politico europeo la responsabilità e l'ipocrisia dei nostri *partner* che a parole hanno sempre professato l'accoglienza, negandola spesso nei fatti. Successivamente, siamo stati testimoni, come non avremmo mai voluto, dell'avverarsi tragico dei più gravi timori su cui avevamo posto l'accento del nostro programma: il crollo del ponte Morandi di Genova ha palesato all'Italia intera le nefaste conseguenze dell'abdicazione dello Stato - e sottolineo abdicazione - dal suo ruolo di regolatore e soprattutto di controllore, di controllore, mettendo inoltre in luce tutte le criticità di un modello di concessioni autostradali promosso, o comunque avallato, dai Governi precedenti, vergognosamente sbilanciato

Abbiamo affrontato la questione con il massimo impegno, su più fronti. Innanzitutto abbiamo pubblicato per la prima volta - ebbene sì - tutti i piani finanziari dei contratti dei concessionari autostradali che contengono - signori miei - quei meccanismi che hanno permesso ai concessionari quegli immani extra profitti. Una trasparenza in nome della correttezza del mercato e della consapevolezza dei cittadini che si attendeva da tanti anni e che non si era mai vista prima. In seconda battuta, in risposta alla tragedia, abbiamo messo in campo soluzioni celeri e concrete, avviando la ricostruzione del ponte senza l'intervento del concessionario. Vi ricorderete che avevamo detto che colui che lo stava gestendo, e non lo aveva manutenuto come avrebbe dovuto, non l'avrebbe mai ricostruito, e L-SP-PSd'Az).* Questa promessa l'abbiamo mantenuta. Ho avuto la fortuna di incontrare tante delle famiglie degli sfollati di Genova

Quando mai si è visto, in Italia, in così poco tempo, a seguito di una tragedia come quella o ad essa simile, un intervento così veloce, immediato ed efficace da parte dello Stato? Anche qui - ripeto - lo avevamo detto e l'abbiamo fatto. Dall'analisi dei piani economici delle concessionarie, finalmente del tutto pubblici, abbiamo inoltre constatato che gli investimenti sostenuti, la manutenzione effettuata e i servizi erogati non erano in linea con le tariffe pagate dai cittadini che passavano al casello e all'inizio dell'anno, per la prima volta, abbiamo bloccato il 90 per cento degli aumenti dei pedaggi autostradali.

che consentirà all'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) di limitare in futuro gli aumenti delle tariffe che potranno addirittura scendere. Ebbene sì: abbiamo bloccato al primo gennaio il 90 per cento degli aumenti e in futuro, alla scadenza del piano economico-finanziario regolatore quinquennale,

a ben vedere, di misure che hanno effetti a lungo termine, niente affatto legate a un orizzonte politico di breve periodo. Ma, siccome con noi lo Stato torna a fare lo Stato, abbiamo ripreso dopo anni a inviare i tecnici del Ministero a fare i sopralluoghi, ad andare sui luoghi a controllare le infrastrutture

fermi da anni o addirittura da decenni - ebbene sì, fermi da anni o addirittura da decenni - e noi stiamo lavorando per sbloccarli. Ne cito a titolo di esempio solo alcuni che abbiamo già sbloccato o stiamo sbloccando: autostrada Asti-Cuneo,

Oltre a questo, stiamo lavorando per migliorare il progetto del passante di Bologna - ieri ho incontrato le autorità locali insieme ai concessionari

Nel contratto di Governo si legge testualmente che «con riguardo alla Linea ad alta velocità Torino-Lione, ci impegniamo a ridiscuterne integralmente il progetto nell'applicazione dell'accordo tra Italia e Francia». Questo impegno è stato la stella polare della mia azione sul *dossier* negli ultimi mesi. Si tratta di un obiettivo che nessuno ragionevolmente potrebbe contestare se si uscisse dalla sterile polemica e si considerasse anche solo la sproporzione

contro l'interesse nazionale. E mi fermo a questo punto senza andare nello specifico. La ridiscussione è un dovere assunto dal Governo in Parlamento fin dalla sua nascita e ribadito testualmente attraverso due distinte mozioni; la prima appena un mese fa alla Camera dei deputati e la seconda solo due settimane fa al Senato della Repubblica. Ho agito totalmente in coerenza e trasparenza, come andrò brevemente a spiegare, evidenziando: lo strumento individuato all'indomani dell'avvio dell'attività di Governo per la ridiscussione dell'opera, come da contratto di Governo, alla base del nostro impegno è stato quello di una nuova analisi costi-benefici che fosse svolta - finalmente, aggiungerei - da un soggetto diverso dal promotore dell'opera o da un soggetto da esso commissionato, a differenza quindi di quanto avvenuto in precedenza; che la composizione del gruppo di lavoro facente parte della struttura tecnica di missione del MIT è stata resa nota fin dallo scorso settembre; in terzo luogo che gli esperti individuati in questo gruppo di lavoro sono riconosciuti a livello internazionale per le loro competenze nell'ambito dell'analisi costi-benefici e nell'ambito dell'economia e ingegneria dei trasporti. Fin dall'avvio dell'analisi costi-benefici è stato affermato pubblicamente che il lavoro è funzionale non all'assunzione di una decisione, ma come contributo alla ridiscussione del progetto. Per consentire il completamento del complesso lavoro di analisi nel rispetto degli accordi con la Francia, come previsto dall'impegno, ho interloquito con la mia omologa francese e ricordato più volte come, all'indomani dell'insediamento del nuovo Governo francese nel 2017, sia stata designata una commissione di esperti per la ridefinizione delle priorità del Paese in ambito di infrastrutture e trasporti. Lo stesso Ministro francese dell'economia ha parlato del progetto in questione come di un investimento ingente, ritenendo del tutto legittimo che il Governo italiano abbia deciso di approfondire nuovamente se possa essere profittevole. Nell'ambito dell'interlocuzione con il Ministro francese è stata condivisa la scelta di rinviare alcuni atti procedimentali relativi all'opera, in attesa delle risultanze dell'analisi costi-benefici, a condizione che queste fossero preventivamente condivise con la Francia e con la Commissione europea. Da lì scaturisce l'esigenza di un confronto preliminare con il nostro *partner* nel progetto e con Bruxelles. Andando avanti sui punti specifici relativi al TAV, ho reso noti questi passaggi e ho proceduto nel senso indicato non appena l'analisi costi-benefici del gruppo di lavoro della Struttura di missione è stata completata. Proseguendo, gli stessi risultati sono stati successivamente e rapidamente inviati al Parlamento, pubblicati sul sito del Ministero e posti alla base della successiva ridiscussione del progetto in seno al Governo. Da ultimo, è stata avviata un'ulteriore fase del procedimento, nel corso della quale il Governo italiano potrà ridiscutere il progetto con l'Esecutivo francese e in sede europea. La condizione per questa ulteriore fase è stata che essa non dovrà comportare ulteriori oneri per lo Stato italiano in caso di recesso. Tutti i passaggi che ho elencato sono stati resi noti tanto al Parlamento quanto all'opinione pubblica, e rientrano evidentemente nell'impegno assunto con il contratto di Governo.

ma ben quattro scenari differenti. In risposta a chi ci accusa di coltivare un atteggiamento pregiudiziale rispetto all'opera, sottolineo che uno degli scenari ha come base

Su questo scenario è stato persino ipotizzato nell'analisi il risparmio derivante dalla cosiddetta *project review*, la quale - lo ricordo - a differenza di quanto affermato dalle opposizioni, risulta essere stata solo oggetto di un'informativa del MIT al

sta introducendo - con assoluta determinazione - alcune misure che velocizzano tantissimi cantieri, e al tempo stesso sta ponendo al centro della sua azione il cittadino che viaggia e l'imprenditore che si muove per lavoro. Ho parlato delle tariffe autostradali. Molti di coloro che hanno depositato le mozioni probabilmente hanno già usufruito del blocco degli aumenti dei pedaggi autostradali che si è avuto all'inizio dell'anno. Ma è importante anche l'impegno per la riforma del codice della strada, che mette al centro la sicurezza e la sostenibilità ambientale, a partire dalla difesa di pedoni, ciclisti e utenti cosiddetti deboli, che, al contrario, vanno percepiti come un'opportunità,

del nostro decreto ministeriale che finalmente obbligherà tutti i gestori delle strade a installare le barriere salva motociclisti. preferisco concludere dando la notizia di un'importantissima misura che a breve porterà un risparmio in termini di tempo e denaro per tutti i cittadini, ossia la portabilità della targa quando si cambia auto: un fatto normale - mi pare di sì e dei trasporti*. Si tratta di una di quelle innovazioni che avvicinano il mio Ministero alla vita di tutti e di cui vado fiero. Gli attacchi che mi sono stati rivolti, tutti concentrati sulla mia persona, e casualmente partiti quando abbiamo messo in discussione il sistema di gestione delle concessioni autostradali...

attacchi rappresentano la migliore prova dell'inconsistenza degli argomenti usati contro il mio operato.

Signor Presidente, gentili colleghi, come sapete, Fratelli d'Italia è sempre stato contrario alle mozioni di sfiducia, perché crediamo che le responsabilità siano dell'intero Governo. Il Governo è un organo collegiale per cui, anche questa volta, noi non abbiamo presentato la mozione di sfiducia, proprio per ciò che ho appena Tuttavia, le devo dire, ministro Toninelli, che in questi nove mesi lei ha dimostrato tutta la sua incapacità. E devo anche sottolineare che mi è dispiaciuto molto vedere un Ministro del MoVimento 5 Stelle che, per la replica, arriva in Aula con un discorso già scritto dagli uffici. Quindi, questo mi fa capire che ha poco rispetto per la democrazia, perché non ha ascoltato gli interventi dei colleghi

vorrei fare un paragone con il calcio che, magari, per lei è più facile comprendere. Quando un allenatore di una squadra di calcio gioca tutte le partite di un campionato e ogni domenica torna a casa con una sonora sconfitta, sonora sconfitta, alla fine viene esonerato o, comunque, capisce che non è il proprio mestiere. Ecco, signor Ministro, le dobbiamo dire con franchezza che questo non è il suo mestiere. lei ora guida non può essere da lei rappresentato: un Ministero così importante, quello delle infrastrutture e trasporti. Purtroppo, devo anche ricordare che il fondatore del suo movimento politico, Beppe Grillo, molte volte ha detto che si tratta di ragazzi e bisogna avere pazienza. No, signor Ministro, sono gli italiani che non possono avere pazienza. Purtroppo, è un lusso che gli italiani non si possono permettere. poi tornare a un'altra parola, che è stata un mantra di tutto il MoVimento 5 Stelle, che è il merito. Voi avete sempre parlato di merito. Dovrebbe farci capire, allora, qual è il merito per il quale lei sta seduto su quella poltrona; qual è il suo *curriculum*; quale esperienze lei ha fatto prima di diventare Ministro delle infrastrutture; qual è il suo apprendistato. Vede, noi non crediamo che l'apprendistato si possa svolgere facendo i Vice *Premier*, i sindaci

che nella memoria degli italiani lei - sì - sarà ricordato, signor Ministro, ma ciò avverrà per molte delle sue *gaffe* che hanno fatto male alla nostra Nazione.

Non so se adesso ha capito che quel tunnel non è mai stato fatto e, se sarà fatto, sarà comunque solo ferroviario. Nella memoria, gli italiani ricorderanno molto bene quando lei, in un'intervista al TG2 Motori, disse

comprare per la sua famiglia un SUV alimentato a diesel? Nella memoria gli italiani ricorderanno, inoltre,

sarà socia del suo Governo in Alitalia. Ricordo che lei li voleva cacciare dalla nostra Nazione perché sanguinari. Dovrà rispondere in questo Parlamento, in quest'Aula,

più rimane seduto su quella poltrona, più i nostri consensi aumentano e i vostri diminuiscono, signor Ministro. Ma noi siamo patrioti, vogliamo il bene della nostra Nazione, vogliamo il bene dell'Italia. Pertanto, crediamo che lei sia pagato per fare le infrastrutture e che gli italiani non la vogliano pagare per non farle. Noi vogliamo più TAV, più alta velocità, dalle Alpi alla Sicilia. Noi vogliamo financo il ponte sullo Stretto di Messina. Noi vogliamo un Ministro che non dica

che anche lei abbia una coscienza e un cuore. Oggi non avrebbe dovuto aspettare una mozione di sfiducia, che - glielo dico onestamente - è un metodo che forse la rafforzerà, perché oggi saranno tutti coesi intorno a lei,

però, signor Ministro, se ha un cuore, si metta una mano sulla coscienza e vada a casa, per il bene dell'Italia e degli italiani. Per tutto questo, il Gruppo Fratelli d'Italia voterà a favore della mozione di sfiducia.

*(PD)*. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, signor Primo Ministro, ministro Toninelli, quello di oggi, dal nostro punto di vista, è un passaggio delicato e importante. Siamo arrivati a presentare una mozione di sfiducia ritenendola l'unico atto possibile per creare le condizioni affinché il Governo torni a lavorare nell'interesse del nostro Paese. sostenuto le nostre tesi, provato a convincervi e - a nostro avviso - prodotto ragioni sufficienti per modificare il suo comportamento e le sue priorità, signor Ministro. Ma lei, con pervicacia e determinazione, è andato avanti sulla sua strada, che porta danno al nostro Paese e alla nostra comunità nazionale. Non ci permettiamo di impostare il ragionamento su questioni personali, come lei giustamente ha denunciato

capire, insieme al Governo e alle forze di maggioranza, i danni che lei, signor Ministro, sta provocando al nostro Paese.

Sono tante le decine di miliardi che aspettano di essere investite e appartengono non a lei, signor Ministro, ma al nostro Paese e alla nostra comunità nazionale:

Il suo intervento, se mi posso permettere, ha rafforzato la nostra convinzione sull'impossibilità che lei continui a svolgere l'importante funzione di Ministro dei trasporti e delle infrastrutture

ma per le sue scelte strategiche contrarie al nostro Paese: questo è il punto. Lei, con metodo e determinazione, ha convinto il Presidente del Consiglio e il Governo tutto a lavorare affinché il nostro Paese fosse bloccato e tante opere pubbliche, già avviate, fossero bloccate su tutto il territorio nazionale, andando contro il nostro futuro e la garanzia del futuro di modernizzare un'Italia che ha bisogno di essere modernizzata e avrebbe le condizioni

dalla parte di quelli che volevano picchiare la polizia e continuate a farlo in Francia perché non avete più il coraggio e la possibilità di farlo in Italia. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Oggi vivete quindi un momento di difficoltà. Qual è allora la sua soluzione signor Ministro?

possa annunciare al Paese che finalmente la TAV è bloccata e finché ci sarà il MoVimento 5 Stelle al Governo essa non andrà avanti. Lo stesso giorno,

interno e verso l'Europa: questo è inammissibile. Questo tipo di comportamento non lo possiamo più accettare. Un Governo deve avere una voce, deve avere un programma, deve fare dei provvedimenti: non può continuare a prendere in giro un Paese intero e lei lo sta facendo insieme ai suoi colleghi. Non è accettabile. Lei si è inventato una commissione, dandogli un mandato in maniera quasi formale, prima che fosse costituita, andando a verificare se le conclusioni sarebbero state quelle che lei stesso avrebbe auspicato. Lei ha sottoposto il Paese a una farsa continua,

che avrebbe ottenuto sulla questione dell'immigrazione. L'unico risultato che ha ottenuto sulla questione dell'immigrazione è aver delegato al Ministro dell'interno le sue funzioni, e questo e questo lo ha certificato ieri lei con il suo partito salvando il ministro Salvini da un processo che era legittimo, auspicabile e un segnale di trasparenza per il nostro Paese e per l'opinione pubblica. *(Applausi dal Gruppo Vede, signor Ministro, purtroppo - lo dico per lei - non siamo soli a criticarla. Nei corridoi dei Palazzi dovrebbe sentire i suoi colleghi di maggioranza che non sono intervenuti in discussione generale: i Ministri della Lega che oggi non sono presenti a supportarla. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Signor Ministro, prenda atto di questa situazione. Abbia il coraggio di avere coscienza della situazione nella quale ha portato il Governo e il Paese, bloccandoci e mettendoci sul fronte del ridicolo, impedendoci di fare legittime battaglie di cofinanziamenti europei per far ripartire il nostro Paese. Signor Ministro, lei si ricorda come ha cominciato? Con l'intervista di un Sottosegretario in televisione che non sapeva chi era il suo Ministro.

Sarà un dato casuale? Signor Ministro, se lo domandi. Riteniamo che ci voglia un gesto di responsabilità, per certi versi anche un gesto autorevole da parte sua e con forza, perché abbiamo capito che lei non cambierà la direzione: non lavorerà per il Passante di Firenze, non lavorerà per la TAV, non lavorerà per gli interventi sui porti, non lavorerà per migliorare la viabilità nel nostro territorio e non lavorerà per sbloccare 27 miliardi di euro che le abbiamo lasciato. Gruppo PD)*. Non lavorerà per far ripartire la nostra economia, per mettersi in contatto e in rapporto con le amministrazioni locali e regionali per sviluppare un grande progetto di rilancio del sistema Paese. Lei è contro tutto questo e ce lo ha dimostrato. Su Genova, signor Ministro, lei ha una colpa che forse è la più grave di tutte: ha provato ad approfittare di una tremenda disgrazia che ha colpito il nostro Paese

incomprensibile e inaccettabile per ognuno di noi. Signor Ministro, lei deve fare una riflessione: sarebbe stato auspicabile un suo passo indietro, una presa d'atto,

Gruppo PD)*. Lei protesta sempre quando gli altri sforano, ma non guarda quello che fa il suo Gruppo che sfora sempre ed io non interrompo

mi faccia parlare. Su questo tema torneremo volentieri in Conferenza dei Capigruppo, perché l'atteggiamento della Presidenza è francamente inaccettabile. l'atteggiamento delle forze di maggioranza nei suoi confronti è evidente; lo si comprende anche visivamente. L'unico motivo per il quale la Lega voterà contro la contro la nostra mozione di sfiducia è perché c'è stato lo scambio nella giornata di ieri, perché voi, rinnegando i vostri princìpi, avete voluto salvare Salvini da un legittimo processo.

Signor Presidente, concludo il mio intervento dicendo che il Gruppo Partito Democratico voterà entrambe le mozioni di sfiducia al ministro Toninelli e io desidero significare la nostra preoccupazione per il Paese consegnando al Ministro l'elenco delle 600 opere che lui ha bloccato, mettendo in ginocchio il nostro Paese, assumendosi e il Governo che rappresenta una grave responsabilità per oggi e per il domani dell'Italia. *(Molti

Tutto ciò a che aiuta a compattare il Governo sarà sempre da noi benvenuto e benvoluto.

un clima di tolleranza e di convivenza pacifica nei confronti dell'immigrazione legale, bisogna essere altrettanto intransigenti nei confronti di quella illegale ed è quello che sia il ministro Salvini che lei invece avete portato avanti in seno

il Ministro doveva seguire; ed è stato seguito con tutto il Dicastero in maniera impeccabile, perché adesso è iniziata la demolizione e i tempi di ricostruzione saranno rispettati. Questa sarebbe già una grandissima novità e un grandissimo cambiamento nel panorama politico italiano in cui sui tempi di realizzazione delle opere siamo purtroppo - ahimè - un po' deficitari. *(Applausi dal mi sottraggo alla famosa questione della TAV o di altre infrastrutture. Però, scusate, adesso lo dico perché le cose poi bisogna ricordarle tutte: che arrivi da una parte della minoranza questa questa volontà di fare a tutti i costi i campioni sul tema delle infrastrutture e delle opere pubbliche sinceramente a me crea qualche problema, ricordando quello che avete fatto in passato. Infatti

La stessa cosa, sempre sulle infrastrutture, la possiamo andare a recuperare con la finanziaria del 2017, e vi dico anche il numero del comma: il 466. atteggiamento, indubbiamente ossequioso nei confronti dei vincoli europei, non ve lo consentiva - avete bloccato 16 miliardi di risorse di cui gli enti locali disponevano e che potevano usare subito per fare gli investimenti. E oggi venite qui a dare lezioni a noi sulle infrastrutture? Ma per favore, un minimo di dignità e di rispetto anche in merito a quello che avete fatto voi al Governo! Invece noi - visto che poi la Consulta ha bocciato quel comma - le risorse le abbiamo sbloccate, tanto è vero che i tanti piccoli cantieri cominciano a partire sui territori. È bastata una circolare; sono bastati degli interventi nella manovra di bilancio; è bastato alzare il tetto di spesa per evitare i famosi bandi rispetto a quel codice degli appalti farraginoso che ha bloccato tante opere e che avete realizzato voi! Come si fa a prendersela con il ministro Toninelli, me lo volete spiegare, quando la maggior parte delle opere oggi ferme sono responsabilità di una cattiva gestione fatta negli anni passati? Invece noi abbiamo sbloccato queste opere, le abbiamo avviate, anche perché abbiamo una strategia un po' diversa rispetto al passato. Sappiamo infatti che non sono importanti solo

perché è caduto un ponte! Guardiamo le responsabilità. Se non facciamo la manutenzione, la responsabilità è tutta nostra, quindi è necessario fare queste opere ed è necessario fare ciò di cui il Paese ha bisogno; quindi sistemare quello che c'è. Poi si faranno anche le grandi opere; certo, abbiamo chiesto di sbloccarle e così sarà. Però non possiamo pensare che la responsabilità di questo Governo sia quella di avere bloccato: non abbiamo bloccato nulla, anzi stiamo andando nella direzione giusta, visto che proprio ieri il Governo ha varato il famoso decreto-legge sblocca-cantieri, che darà un'ulteriore accelerata in questa direzione. Alla luce di questo, il nostro voto non è un no alla mozione di sfiducia, ma un sì alla fiducia che oggi voteremo nei confronti del ministro Toninelli e di tutto il Governo. *(Molti

e mi ha fatto capire che la politica è proprio un'arte, perché se lui riesce a difendere Toninelli, vuol dire che è proprio un fuoriclasse. *(Applausi dal per la politica dei migranti: lo ha ringraziato perché il ministro Toninelli è stato di fatto destituito dal suo ruolo da Salvini. È per questo che l'ha ringraziato *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*: perché non ha fatto il Ministro dei trasporti e delle infrastrutture

in imbarazzo, perché quando un partito ti chiede di intervenire in dichiarazione di voto è un grande onore per ognuno di noi. Per me invece è motivo di imbarazzo in questo caso, per la storia del mio partito, signor Presidente. Infatti, il mio partito - ha detto bene la collega prima di me non ha mai fatto una mozione di sfiducia; mai, perché noi siamo garantisti a prescindere. E sono imbarazzo per la mia storia personale - mi permetta - perché ho avuto l'onore e l'onere di fare il Presidente di una Regione, quindi può immaginare quante volte hanno chiesto le mie dimissioni. Quindi c'è un grande imbarazzo. Noi chiediamo le dimissioni del ministro Toninelli non per svariati altri motivi, di cui abbiamo discusso qui (perché magari il parente o l'affine ha fatto un regalo

passata esperienza: ha fatto il carabiniere, l'assicuratore e ha fatto un buon lavoro - gliene do atto - nella passata legislatura in Commissione affari costituzionali. Questo era il suo ruolo, probabilmente, non certo quello di Ministro delle Ma l'inesperienza - noi abbiamo altri casi di personalità che sono lì sedute tra i Ministri - è normale: tutti abbiamo avuto inesperienza quando abbiamo ricoperto ruoli importanti. Ognuno di noi in quest'Aula parla

Così ha fatto Conte, così ha fatto Di Maio, così hanno fatto altri: studiano. Poi non siamo d'accordo, ma almeno studiano, approfondiscono i *dossier*. Lei, signor Ministro, assolutamente mai. C'è un elenco infinito di questioni che lei non ha approfondito. Ad esempio, parlando di Genova,

polifunzionale, vivibile, percorribile, transitabile? È un ponte alto cinquanta metri. Se lei avesse approfondito saprebbe, signor Ministro, che le autostrade da lei tanto vituperate

Nessuno ce l'ha con lei. Guardi che i comici che la prendono in giro non ce l'hanno con lei: è lei che ce l'ha con noi. *(Applausi dai Gruppi Se la Confindustria dice che lei è una vergogna, se il direttore di un giornale come «La Stampa» dice che lei straparla, se Grillo dice di non sparare su Toninelli perché è come sparare sulla Croce Rossa, non sono io, non è Forza Italia, non è il PD.

una dietro. Prima di andare a fare un'intervista anche io mi preparo come tutti, ma non è pensabile che il Ministro possa aver detto e fatto ciò che poi ha detto e fatto, cioè comprare una macchina *diesel*.

Sono andato a vedere (mi intendo di queste cose): la Jeep Compass che ha comprato il Ministro costa circa, a seconda delle versioni, dai 25.000 ai 30.000 euro. Con gli stessi soldi, o con meno, avrebbe potuto comprare

un dramma per il settore dell'*automotive*: chiuderanno decine e decine di concessionarie. Oggi è il 21

Senatore Patuanelli, lei sa benissimo che l'intervento che ha fatto il senatore Airola mentre il senatore Biasotti faceva la sua dichiarazione di voto è

Presidente, potrei impiegare veramente poco tempo per fare la mia dichiarazione di voto perché il Ministro Toninelli ha esplicitato in modo chiaro qual è stata l'attività del Governo, del suo Ministero e dei Sottosegretari ed io, che ho la fortuna di lavorare molto spesso, essendo anche membro dell'8a Commissione, assieme al suo Ministero e al e al Ministro, guardo invece all'impegno e alla capacità di studiare e di approfondire i *dossier*, i tanti *dossier* aperti che abbiamo trovato in questo Paese e che oggi dobbiamo portare avanti. Mi sembra del tutto evidente che la discussione che si è svolta in quest'Aula rispetto alle due mozioni di sfiducia che segnano l'idillio che continua tra Forza Italia e il Partito Democratico, un matrimonio che ci continua a far felici... In questa discussione si è parlato di grandi opere e di infrastrutture, in sostanza si è parlato di una concezione di sviluppo che è in realtà è una concezione sbagliata di sviluppo. Il fare opere tanto per farle è una concezione sbagliata. Ho sentito parlare di decrescita felice perché forse, questo sì per ignoranza, non si conosce il concetto di economia circolare, PATUANELLI *(M5S)*. Io credo che oggi non si possa contemporaneamente parlare di quelle grandi opere e poi applaudire Greta Thunberg quando fa le sue manifestazioni, perché o si rispetta l'ambiente o si parla di opere inutili. Le due cose assieme non si possono fare. La prima idea di questo Governo è di far spendere i soldi dei nostri cittadini con rispetto, analizzando gli effetti che una determinata spesa ha sul pubblico e su tutti gli investimenti per cui fare analisi costi-benefici con enti terzi e non con i proponenti è un elemento essenziale per vedere come spendere i soldi degli italiani; altrimenti continuiamo continuiamo a fare cose che non servono al Paese e continuiamo ad accrescere il debito pubblico. Questo è quello che è successo: abbiamo fatto opere inutili che poi non siamo nemmeno in grado di manutenere, come dimostra in modo evidente il sistema infrastrutturale del Paese che è in condizioni fatiscenti perché non è mai stato speso un centesimo per la giusta manutenzione. Quando si parla di sviluppo si parla sempre di infrastrutture materiali, invece è evidente che questo Governo sta facendo anche un passo molto importante verso l'infrastrutturazione immateriale del Paese, verso le nuove tecnologie, verso lo sviluppo lo sviluppo sostenibile, verso tutte quelle cose che hanno obbligato questo Paese ad essere arretrato rispetto ad altri Paesi europei *(Applausi dai delle nostre imprese di fare un salto tecnologico, che è fondamentale. Noi abbiamo un tessuto imprenditoriale che non è fatto da grandi imprese, ma da un tessuto di piccole, medie e microimprese ed è nella direzione di quel sistema economico che dobbiamo quindi muovere le azioni di Governo. Ha poco senso parlare di opere da 10 miliardi di euro che hanno una ricaduta economica, perché le nostre imprese saranno poco chiamate a realizzare quelle opere. Abbiamo bisogno di fare, come diceva anche il senatore Romeo, tante piccole opere; l'abbiamo fatto con i 400 milioni di euro per i piccoli Comuni *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az)*, sbloccando gli avanzi di amministrazione dei Comuni virtuosi. Queste sono le opere che

un quadro complessivo sul sistema infrastrutturale, non posso esimermi dal parlare «del» TAV; rilevo che non si è neanche in grado di vedere che se un sostantivo è maschile - il treno - l'articolo non può essere femminile. Il TAV non è

L'impegno di questo Esecutivo contrattualizzato nel contratto di Governo, è quello di rivedere integralmente l'opera ed è ciò che il ministro Toninelli, assieme al Presidente del Consiglio, sta facendo giustamente e preliminarmente con la Francia e poi farà con i *partner* europei. Sono certo che la soluzione si troverà, perché mi sembra evidente che alla fine c'è un disegno narrativo che vuole dividere una maggioranza che invece è unita e sta governando molto bene questo Paese. Detto ciò, Presidente, mi sembra evidente che il Gruppo che mi onoro di presiedere voterà convintamente a favore della fiducia al ministro Toninelli e all'operato del Governo. Ho sentito dire da una collega che essere Toninelli oggi, è difficile; io dico che essere Toninelli oggi, è avere la schiena dritta. *(I

votazione delle mozioni, pur considerando corretto da parte del mio Gruppo, nell'attuale situazione,

Infatti ieri, cari colleghi senatori, senza il voto di Fratelli d'Italia e di Forza Italia, il Governo sarebbe caduto non avendo raggiunto il numero prescritto

il suo modo di presiedere, anche per aver stigmatizzato una frase che magari poteva essere battutistica. Ha fatto benissimo, perché è vero, caro collega,

la ringrazio e mi auguro che presto l'Italia possa avere un Governo che non abbia bisogno di soccorsi tricolori per esistere.

i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza. Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello

Ciriani De Bertoldi,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

i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza. Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello Siri).* Invito il senatore Segretario a procedere all'appello,

alle quali risponderanno il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

signor Ministro, l'interrogazione riguarda la chiusura dell'ospedale e del primo soccorso, ad esso ovviamente collegato, di Città della Pieve in Umbria, ma ha un interesse nazionale poiché coinvolge, potenzialmente e indirettamente, tutta la rete ospedaliera dell'emergenza-urgenza, come è facile dedurre dai fatti.

le attività a carattere ospedaliero, compreso il primo soccorso, a Città della Pieve. Il 24 aprile 2017, il Comune di Montegabbione, i cui cittadini fruivano dei servizi soppressi in ragione della vicinanza territoriale, ricorreva al TAR dell'Umbria contro l'azienda unità sanitaria locale Umbria n. 1 e contro la Regione Umbria (come controinteressato) per l'annullamento, previa sospensiva, della citata delibera. Il 7 febbraio 2018 il TAR, con sentenza n. 98/2018, accoglieva il ricorso, in particolare relativamente alla contestata chiusura del pronto soccorso, riconoscendo il supremo interesse al diritto alla salute e ordinandone la riapertura. La Regione ha successivamente fatto ricorso al Consiglio di Stato e, nella sentenza, il Consiglio di Stato entra nel merito della *golden hour*, quell'ora fondamentale, la cosiddetta ora d'oro che determina, in molti casi, la salvezza del paziente appunto, quelle che sono considerate le morti evitabili. Su questo, tutti ritengono che l'ora parta dal momento di intervento dell'ambulanza fino all'arrivo al presidio più vicino. La sentenza, contrariamente, tiene conto del tempo dal momento in cui l'ambulanza è già presente sul luogo dei fatti. Una eventuale interpretazione di questo tipo potrebbe costituire un precedente drammatico, soprattutto per tutte quelle aree di particolare disagio che sono, comunque, riconosciute dal decreto ministeriale n. 70, e per le quali sarebbe possibile intervenire in deroga alle disposizioni del decreto stesso. Quindi, l'interrogazione è volta a conoscere la posizione del Ministro e a sapere se non sia il caso di intervenire sui tavoli ministeriali per dare una versione univoca ed effettiva di come debba essere calcolato il tempo di intervento, che è ovviamente uno degli aspetti fondamentali, non l'unico, ma sicuramente determinante, anche in rapporto ai servizi offerti dai presidi

Signor Presidente, ringrazio il senatore interrogante perché, partendo da un episodio specifico, mi consente di fare chiarezza su una questione più generale, quella relativa agli interventi di emergenza-urgenza, che costituisce davvero un tratto qualificante per misurare l'efficienza del Servizio sanitario nazionale.

nell'ambito dell'assistenza ai traumi, per i quali la tempestività dell'intervento sanitario influisce, senza alcun dubbio, sulle possibilità di sopravvivenza. Occorre precisare che tale concetto, in ogni caso, non si riferisce esclusivamente all'intervallo temporale di sessanta minuti: esso, piuttosto, mira a garantire, più in generale, la migliore tempestività

tra presidi sul territorio, ma va piuttosto parametrato sulla capacità di stabilire un primo contatto del paziente con operatori sanitari qualificati, se del caso anche in ambito preospedaliero. L'organizzazione delle reti tempo-dipendenti, così come previsto dal decreto ministeriale n. 70 del 2015, tiene ovviamente bene in conto tali principi: essa, infatti, definisce il sistema organizzato per la gestione delle emergenze in modo che sia garantita l'integrazione dei sistemi di intervento di emergenza-urgenza con il territorio e con gli ospedali organizzati a diversa complessità assistenziale. La stessa sentenza citata nell'interrogazione, peraltro, riafferma con chiarezza questo principio, in quanto precisa che i tempi di percorrenza debbono essere valutati non solo in relazione ai presidi sul territorio, ma anche in relazione alla dislocazione e alla funzionalità del Fatte queste precisazioni, e ritenuto, dunque, che la sentenza del Consiglio di Stato non imponga la necessità di adottare ulteriori chiarimenti interpretativi, ne deriva che per assicurare davvero la tempestività dell'assistenza nel campo dell'emergenza-urgenza, il compito del Ministero della salute è ben più complesso di quello che deriva dalla mera analisi dei tempi di percorrenza tra presidi sul territorio. Proprio sulla base di questa consapevolezza, intendo, allora, assicurare che il Ministero della salute, attraverso i tavoli di monitoraggio e verifica del è in grado di sviluppare un'azione di controllo e di impulso ai fini del miglioramento di tali reti a livello regionale e dello sviluppo in tutto il territorio nazionale, nonché di analizzare ogni eventuale "fatto nuovo" - sia esso determinato da nuove evidenze scientifiche o da circostanze quali quella rappresentata dall'interrogante - in modo da predisporre ogni conseguente iniziativa che assicuri l'omogeneità dell'assistenza di emergenza-urgenza sul territorio nazionale. PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Briziarelli, il Ministro e mi dichiaro parzialmente soddisfatto. Sono ovviamente soddisfatto per il riconoscimento della valenza nazionale del tema e per tre aspetti in particolare. si riconosce la valenza scientifica della *golden hour*; addirittura si va oltre, dicendo che il tempo di intervento è fondamentale, ma

mi fa piacere la disponibilità, attraverso i tavoli, a valutare il caso di specie e le eventuali novità. In questo senso, vorrei sottolineare che, delle due, l'una: o c'è un'interpretazione, non voglio dire errata, ma parziale, che peraltro, nel fatto di specie, tiene conto di una documentazione da parte della ASL, che fornisce i tempi relativi - ripeto - alla presenza sul posto e non alla partenza, superando quindi anche i tempi di novanta minuti per il raggiungimento degli *hub* e non solo dei sessanta minuti della vicinanza per il primo intervento; oppure i criteri interpretativi sono da cambiare perché in contrasto, di fatto, con i principi costituzionali già riconosciuti dal TAR e che il Consiglio di Stato prende in considerazione, relativamente al diritto supremo alla salute per quanto riguarda l'emergenza-urgenza. Mi riservo, quindi, di fornire al Ministero tutta la documentazione affinché sia esaminata nei tavoli.

Signor Presidente, signor Ministro, faccio una breve premessa: 16.700 medici specialisti in meno nel 2025. Questa è una comunicazione di ieri di ANAAO Assomed, che dimostra che ci sono pochi giovani rispetto ai pensionati e a coloro che chiederanno di andare in pensione anche con quota 100. sicuramente disservizi nel Sistema sanitario nazionale, con grandi criticità soprattutto nelle Regioni Sicilia e Piemonte. Non basteranno quindi i neospecialisti a sostituire chi andrà in pensione e il saldo tra chi entra e chi esce dal 2018 al 2025 si tradurrà in queste enormi cifre. Ora passiamo all'illustrazione di questa nostra interrogazione, che si aggancia palesemente a quanto vi ho appena anticipato. Parliamo dello svolgimento dei tirocini professionalizzanti per i laureati in medicina di cui alla circolare ministeriale n. 9498 del 18 marzo 2019, che è appena stata inviata alle università e indica i tempi per svolgimento e che darà la possibilità di fare gli esami di Stato necessari ad accedere alle scuole di specialità agli studenti iscritti all'anno accademico 2017-2018. non sanno ancora nulla, invece, gli studenti che si laureeranno nell'anno accademico 2018-2019, che andrà da giugno 2019 fino a marzo 2020. Non vi è quindi alcuna certezza di quello che succederà, cosa che creerà inevitabilmente confusione, oltre al fatto che l'esame di ammissione alla scuola di specializzazione il tirocinio, l'esame di Stato e la scuola di specializzazione sono tappe che si devono allineare. Non sappiamo quindi ancora nulla, perché tra l'altro l'esame di ammissione alla scuola di specializzazione è avvenuto con otto mesi di ritardo: solitamente era novembre, mentre quest'anno è andato a finire a luglio 2018, quindi l'anno scorso. Questo disallineamento disallineamento provocherà sicuramente un rallentamento anche dell'ingresso nelle scuole di specialità e quindi creerà un imbuto formativo che purtroppo non farà altro che peggiorare la situazione.

di svolgimento sarà fissata prossimamente con apposita ordinanza di quel Ministero. e in particolare se i quesiti somministrati saranno estratti da un archivio informatico periodicamente aggiornato oppure predisposti da quel Ministero avvalendosi di apposita Commissione nazionale di esperti. Il citato Dicastero, in ogni caso, ha dato ampia assicurazione che l'ordinanza ministeriale in questione verrà adottata in tempi congrui a consentire lo svolgimento della prossima sessione d'esame. Devo però chiarire con decisione che le problematiche connesse alla tempistica dell'indizione della prossima sessione degli esami di Stato, che, come si è detto, è ferma intenzione del MIUR fissare al più presso, non condizioneranno l'accesso al concorso per le scuole di specializzazione di area sanitaria. Ricordo infatti che costituisce requisito di accesso a tale concorso il possesso della laurea magistrale in medicina e chirurgia, mentre quello dell'abilitazione è richiesto solo al momento dell'inizio delle attività didattiche, solitamente previsto per i primi di novembre. Per ciò che riguarda le competenze del Ministero della salute, intendo dare assicurazione che in merito alla problematica relativa alla carenze di medici specialisti, che, come noto, ha già formato oggetto di specifici interventi da parte del Governo, proprio in questi giorni sono in atto le opportune interlocuzioni con i competenti uffici del MIUR, che, ne sono certa, produrranno soluzioni condivise in grado di evitare

Ministro, lei ha perso un'occasione oggi, glielo dico di cuore, perché non è qui per farci un piacere, ma è interrogata ed è suo dovere venire a rispondere alle

gli Uffici hanno ritenuto che il quesito che abbiamo posto fosse un quesito adatto a lei, perché chiedevamo a lei in che modo intenda risolvere il problema. La risposta, Ministro, doveva essere: «aumentando le borse di studio e aumentando i posti».

una ragione: proprio perché non siete stati attenti a far partire le questioni come Governo (in fondo vi assumete sempre le responsabilità come Governo, ce l'avete detto qui in Aula anche ieri; non è mai la responsabilità del singolo, ma sono sempre decisioni governative), si troveranno a fare il tirocinio *post lauream* insieme agli studenti che si stanno ancora preparando per la laurea, quindi *ante lauream*, secondo quella che dovrebbe essere la nuova norma. Ecco qual è l'imbuto su cui lei non ha voluto assolutamente rispondere. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Però ci dovrà dire prima o poi - e lo dovrà dire ai ragazzi - come intende limitare questo sovraffollamento, che significa meno qualità, meno sicurezza e minore possibilità di prepararsi, com'è loro diritto.

Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, l'ultima legge di bilancio ha stabilito che per gli anni 2020-2021 l'accesso delle Regioni all'incremento del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale sia subordinato alla stipula, entro il 31 marzo 2019, del Patto per la salute 2019-2021 che includa misure di programmazione e miglioramento della qualità delle cure e dei servizi erogati e di efficientamento dei costi. Il 13 febbraio 2019 le Regioni hanno elaborato un documento programmatico sui temi principali che dovrebbero caratterizzare il Patto per la salute, chiedendo al Governo di: prevedere una revisione dei meccanismi di controllo dei processi e dei costi, individuando indicatori significativi di risultato sullo stato di salute dei singoli sistemi sanitari regionali, affrontare il tema della *governance* del Sistema sanitario nazionale, dei ruoli e dei rapporti tra gli attori istituzionali coinvolti (quindi Governo, Regioni, AIFA, Agenas, Istituto superiore di sanità) e rimettere al centro dell'azione la formazione e la valorizzazione del capitale umano, prevedendo nuove metodologie di definizione dei fabbisogni organizzativi e formativi coerenti agli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e regionale. Noi condividiamo in pieno, Ministro, la sua visione secondo cui il Sistema sanitario nazionale rappresenti una pietra miliare nello sviluppo e nella coesione sociale del Paese ed è quindi necessario che la sanità sia messa al centro delle azioni e dell'agenda di Governo, per fornire ai cittadini servizi sanitari efficaci, innovativi e qualitativamente adeguati da Nord a Sud, perseguendo la sostenibilità del sistema attraverso l'efficienza dei propri processi programmatori organizzativi e di produzione. È un dato di fatto però che la sanità sia proprio il comparto del settore pubblico che ha visto costantemente scendere il suo livello di finanziamento in proporzione al PIL, scontando anche la volontà dei Governi precedenti di trasferire in capo alle Regioni le difficoltà di sostenere le politiche pubbliche in periodi di crisi finanziaria, nonostante numerosi studi abbiamo indicato, al contrario, come proprio nelle fasi critiche del ciclo economico l'investimento nel settore salute sia in grado di produrre effetti a breve termine e, quindi, contribuire significativamente alla ripresa economica. Alla luce di queste osservazioni le chiediamo, Ministro, quali azioni intenda adottare per implementare il nuovo Patto per la salute 2019-2021, in vista della scadenza del 31 marzo, e come intenda intervenire nel Patto per la salute affinché sia garantito il principio di uguaglianza dei cittadini nell'accesso alle cure

ringrazio davvero gli interroganti, perché mi permettono di illustrare, per quanto sinteticamente, i principi ispiratori dell'azione del Governo nel percorso che porterà - confido quanto prima - all'adozione del prossimo Patto per la salute. Innanzitutto, va detto che le Regioni hanno fornito negli ultimi anni numerose prove di collaborazione istituzionale, giungendo al miglioramento di molti indicatori di efficienza e contribuendo lealmente alle manovre di finanza pubblica. di salute di ogni sistema regionale. Di converso, il mancato rispetto di tali indicatori comporterà la piena responsabilità della Regione e dei suoi organi di Governo. Alle Regioni in difficoltà, in ogni caso, dovranno essere assicurate nuove forme

per programmare correttamente gli interventi sui territori regionali. Concludo con quello che, per molti versi, ritengo il principale fattore qualificante del Patto. In esso, infatti, dovrà tornare al centro la formazione, la qualificazione e la valorizzazione del capitale umano, prevedendo nuove metodologie di definizione dei fabbisogni organizzativi e formativi, nonché la semplificazione dell'accesso dei professionisti e degli operatori al Servizio sanitario nazionale per ottenere un efficace e tempestiva copertura degli stessi fabbisogni che, come sappiamo, risultano essere in grave sofferenza, Su tali ultimi aspetti, peraltro, mi sia consentito di affermare con orgoglio che il Governo, prima e indipendentemente dal prossimo Patto per la salute, come il Parlamento ben sa, tanto ha già fatto e tanto ancora si è impegnato a fare. A conferma di ciò consentitemi di citare, fra le cose già fatte, il piano per l'abbattimento delle liste di attesa, con la destinazione finalmente di considerevoli risorse economiche e soprattutto - la notizia è di oggi - il via libera delle Regioni ad un'ipotesi normativa che superi

Signor Ministro, sono pienamente soddisfatta della sua risposta. Voglio anche sottolineare come il superamento del blocco delle assunzioni, che lei ha appena annunciato e di cui noi abbiamo letto letto proprio oggi, è per noi un segnale di grande speranza, soprattutto perché interesserà anche le Regioni in piano di rientro e noi sappiamo quanto siano proprio queste ad avere più bisogno di assumere personale per raggiungere finalmente i livelli essenziali di assistenza e permettere

dell'odierno *question time* si incentra quindi proprio sulla *flat tax*, o meglio sulle *flat tax*, visto che di più *flat tax* dobbiamo e possiamo parlare alla luce di quanto è successo.

Vede, signor Ministro, voi, la vostra maggioranza e il suo Governo avete venduto come *flat tax* realizzata quella per i lavoratori autonomi inserita nella scorsa legge di bilancio. Vorrei chiederle cosa pensa del fatto che su 4 milioni circa di partite IVA, solo 320.000, quindi poco meno dell'8 per cento, possono usufruire oggi della *flat tax* che voi dite essere stata realizzata per il lavoro autonomo.

con il documento in esame i senatori interroganti, nel richiamare una proposta della passata legislatura volta a introdurre l'applicazione di un'aliquota unica agevolata sugli aumenti retributivi e di reddito aumenti retributivi e di reddito percepiti in misura maggiore rispetto all'anno precedente, chiedono di sapere quali siano gli intendimenti del Governo in ordine all'introduzione di una *flat tax* incrementale estesa all'intera platea dei contribuenti. È opportuno ricordare che la legge di bilancio 2019 ha potenziato e migliorato il regime forfetario. Tutti i soggetti che esercitano attività di impresa, arti o professioni beneficiano di un regime fiscale caratterizzato da forfettizzazione della base imponibile, tassazione sostitutiva di Irpef e IRAP con aliquota del 15 per cento e sono esclusi dal campo di applicazione IVA e godono di significative semplificazioni contabili e in termini di adempimenti. Alla luce delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2019, dal 2020 circa 1,5 milioni di soggetti fruiranno dei suddetti regimi agevolati, ossia una platea di contribuenti che rappresentano circa il 40 per cento della totalità dei soggetti titolari di partita IVA. Si tratta ovviamente dell'avvio di un processo di riforma che è coerente con gli indirizzi contenuti all'interno del contratto di Governo e secondo una logica di attuazione progressiva delle riforme, rese in questo modo compatibili con i vincoli di finanza pubblica. Ciò premesso, sarà in sede di predisposizione della prossima manovra di bilancio, così come avvenuto nella precedente, che potranno essere esplicitate le diverse ipotesi di riforma fiscale addizionali. In detta occasione

come già ho affermato in altre circostanze, che al momento non è stata formulata alcuna stima ufficiale in merito a specifiche proposte di riforma. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze, fin dal luglio scorso (non so prima) sono state condotte molte analisi concernenti varie ipotesi di riforma fiscale. Si tratta di un esercizio di valutazione *ex ante* delle *policy*, che, oltre a riferirsi al contenuto delle misure, riguarda anche gli aggiornamenti dei modelli di microsimulazione. Queste attività sono fondamentali per creare le condizioni e la base conoscitiva utile a stimare l'impatto delle misure di Governo, ma certamente non possono essere utilizzate

l'apertura che lei rivolge al nostro disegno di legge e l'intenzione del Governo di valutare al meglio una misura affinché possa essere realmente applicata a tutti i contribuenti tutti i contribuenti e - ribadisco - possa davvero dare uno stimolo a chi vuole lavorare di più, a chi vuole produrre di più e quindi essere ricompensato con una più bassa tassazione sul reddito incrementale, e contemporaneamente rendere sconveniente, anche da un punto di vista monetario, il sommerso, quindi il nero. Apprezzo questo suo intendimento e questa sua apertura. Noi siamo disponibili ed aperti a ogni collaborazione nei confronti della maggioranza, laddove ci si muova nell'ottica di stimolare davvero l'economia e di ridurre quindi una pressione fiscale oggi inaccettabile. Naturalmente, essendo alle porte il DEF, auspichiamo, come Fratelli d'Italia, che il Governo possa dirci già nel DEF qualcosa di più, entrando più nel merito dei progetti che saranno poi tradotti nelle leggi di bilancio per il 2020. Quindi, signor Ministro, apprezzo la sua apertura, ma soprattutto auspico davvero che da parte della maggioranza e dell'intero Parlamento ci sia al più presto una condivisione di questi progetti per la crescita del nostro Paese. apre una nuova finestra"). Salutiamo studenti e docenti del Liceo scientifico «Enrico Fermi» di Massa, che stanno assistendo ai nostri lavori.

Evidentemente la *flat tax* ha un costo, che era stimato in 50 miliardi di euro, da fronteggiare, soprattutto nel primo e nel secondo anno (a seconda delle proiezioni, dal terzo anno dovrebbe dare dei risultati positivi), con la riduzione degli sconti fiscali maggior controllo della spesa (ci sta ancora). Attenzione poi al debito pubblico e soprattutto allo *spread*: io dico che sarebbe opportuno evitare dichiarazioni troppo facili che possono spostare di centinaia di milioni e anche di miliardi di euro il calcolo degli interessi. recupero evasione per emersione. Dalla *flat tax* sarebbero venuti - lei ha riconosciuto - più investimenti e più consumi. Per ora si è iniziato con un numero limitato, come diceva il collega, con un'aliquota al 15 per cento. Il ministro Salvini ha detto che si farà per tutti al 15

Ieri il sottosegretario Siri ha dichiarato che si farebbe per nuclei familiari fino a 50.000 euro e che costa 12 miliardi di euro. C'è qualche disaccordo tra alleati? Ci sono delle diverse vedute?

di conoscere quali siano gli intendimenti del Governo in ordine all'introduzione di una *flat tax*, a quanto ammonterebbero i costi e in che modo sarebbero reperite le risorse necessarie. Rispondo scusandomi fin dall'inizio di alcune inevitabili ripetizioni. Innanzitutto voglio ricordare che la *flat tax* è da declinare al presente e non al futuro, perché con la legge di bilancio per il 2019 il Governo è intervenuto, in maniera graduale, per ridurre la pressione fiscale relativa al reddito delle persone fisiche e delle imprese. La misura prevede che gli esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo possano optare per un regime agevolato, con aliquota al 15 per cento, insieme ad altre semplificazioni fiscali. la ripetizione: ricordo sempre che, alla luce di queste novità, circa il 40 per cento della totalità dei soggetti titolari di partita IVA fruirà dei suddetti regimi agevolati. Queste misure fiscali già adottate sono parte dell'azione di riforma che il Governo intende proseguire durante tutto l'arco della legislatura. Tale azione si ispira ad una logica di progressiva attuazione del programma di Governo, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. In sede di predisposizione della prossima manovra di bilancio, saranno valutate altre ipotesi di riforma fiscale, ispirate evidentemente

forse ormai inutile, per precisare che non è stata formulata alcuna stima circa l'impatto di una possibile estensione della *flat tax,* aproposito delle

per essere in grado di valutare ogni ipotesi concreta di riforma, nel momento in cui questa si pone concretamente all'attenzione del decisore politico. Quindi, utilizzare risultati ed esercizi

Avrei adottato volentieri la teoria dell'*helicopter money*, che è tramontata subito, ma era simpatica: buttare soldi dall'elicottero, così chi li prende prima li può spendere e fa aumentare i consumi.

e del turismo* - Premesso che: uno dei prodotti italiani a denominazione tra i più famosi nel mondo è il Pecorino romano Dop, la cui zona di produzione comprende il territorio del Lazio e quello della Sardegna, con 15.000 aziende zootecniche su 50.000 complessive. Conseguentemente alla sovrapproduzione e ad un calo dei consumi, in questi ultimi mesi si sono avuti risvolti sui prezzi di acquisto, acquisto, applicati non solo dalle imprese, ma anche dalle cooperative di trasformazione degli stessi allevatori. Il prezzo del latte ovino, che a inizio 2018 era pari a 85 centesimi al litro,

Il prezzo del formaggio pecorino all'ingrosso è sceso, infatti, tra il 2017 e il 2018 da 7,7 euro al chilogrammo a 5,2 euro al chilogrammo, mentre i prezzi nella grande distribuzione organizzata sono sostanzialmente elevati (18,90 euro al chilo presso la Conad). In un momento in cui pastori e allevatori fanno i salti mortali per sopravvivere, il pecorino romano viene addirittura importato dalla Romania e finanziato dal Governo italiano, per essere stagionato poi in Sardegna e diventare, secondo le assurde norme del codice doganale, prodotto italiano. Questo *modus operandi* causa il deprezzamento della materia prima e danneggia uno dei prodotti più famosi nel mondo come, appunto, il pecorino romano. Tra le industrie più note vi è quella dei fratelli Pinna. Tale azienda ha avuto un contenzioso giudiziario nel 2010. L'associazione degli allevatori aveva diramato un comunicato contro i formaggi prodotti dall'azienda in Romania che, con nomi e bandiera italiana sulla confezione, potevano trarre in inganno i consumatori. Chiedo, pertanto, al Ministro di sapere se l'assegnazione di risorse a caseifici che hanno provocato eccedenze sia compatibile sia con le regole della concorrenza dell'Unione europea, che con le norme sulla concorrenza previste dall'Italia e non configuri aiuti di Stato; se il Ministro voglia chiedere all'*Antitrust* di accertare se è vero che nel periodo intercorrente tra il mese di marzo e aprile 2016 i caseifici abbiano deciso un abbassamento del prezzo in maniera allineata comunicandolo agli allevatori

recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari. La finalità di tale provvedimento risiede nella necessità e urgenza di sviluppare, oltre che per il settore olivicolo, oleario e agrumicolo, anche per quello ovino-caprino un piano di interventi per il recupero della capacità produttiva e per sostenere concretamente le imprese agroalimentari. Per quanto attiene nello specifico alle misure di sostegno del settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino, il decreto istituisce un fondo dedicato con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per l'anno 2019 finalizzato a favorire la qualità e la competitività del latte ovino attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, l'adozione di misure temporanee di regolazione della produzione, compreso lo stoccaggio privato dei formaggi ovini a denominazione di origine protetta (le cosiddette DOP),

SA.42821-contratti di filiera e di distretto, autorizzato dalla Commissione europea o, in alternativa, a ogni singolo produttore nel rispetto del regime *de minimis*. Allo scopo di assicurare un accurato monitoraggio delle produzioni lattiero-casearie realizzate sul territorio nazionale si introduce l'obbligo di registrazione della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti caseari a base di latte importati dai Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi. Riguardo poi alla segnalata indagine da parte dell'Autorità garante della concorrenza in merito al comportamento tenuto dai caseifici aderenti al consorzio del pecorino romano DOP in relazione alla determinazione del prezzo del latte pagato agli agricoltori, segnalo che il Governo, in linea con il Parlamento, sta seguendo con attenzione l'*iter* già avviato dalla predetta autorità. In tale contesto mi preme evidenziare l'impegno assunto per valutare un accordo per l'adozione di disciplinari che prevedano sanzioni efficaci per il caso di mancato rispetto dei quantitativi di produzione del pecorino romano e di qualunque altro prodotto lattiero-caseario DOP che siano causa del deprezzamento della materia prima. In ogni caso, il pecorino romano DOP beneficia di un piano per la regolazione dell'offerta predisposto dal consorzio per il triennio 2016-2018 e prorogato proprio pochi giorni fa fino a luglio 2019 dal sottoscritto, che prevede misure disincentivanti per i produttori di pecorino che non rispettino le quote di produzione loro assegnate. Quanto poi alla norma del codice doganale che consente di ritenere originario di uno Stato membro un prodotto che ha avuto soltanto l'ultima fase di trasformazione eseguita in quello Stato, faccio presente che trattasi di disposizione a carattere orizzontale, non specifica per il pecorino romano. In ogni caso la sua eventuale modifica o soppressione non rientra nelle competenze del mio Ministero. Concordo, tuttavia, sull'opportunità di ulteriori approfondimenti tesi ad individuare eventuali condizioni che consentano di superare tali criticità.

cassette da sei a cassette da tre e diventavano prodotto nazionale. È un tema che dovrebbe impegnare l'Unione europea a rivedere questa norma doganale assurda, così come è importante,

al quale chiedo se si vuole scongiurare la soppressione del tribunale di Vasto e garantire alla collettività e ai territori interessati la permanenza di uffici a presidio di diritti e garanzie irrinunciabili. Contestualmente approfitto per auspicare anche una risposta scritta all'interrogazione

Un caso in cui ho rilevato, tra le altre cose, il mancato trasferimento in una struttura idonea e nessuna decisione di cura in conseguenza ai colloqui individuali con educatori professionali (psicologi e psichiatri) che non potevano non sapere dei disagi del detenuto. La ringrazio della sua eventuale intercessione in merito a questi solleciti.